dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

sulla materia dell'ordinamento professionale riproponesse antichissime questioni, dibattiti ed opzioni con riferimento all'organizzazione e alla disciplina dell'avvocatura. Così come era inevitabilmente scontato che accadesse con ricaduta sull'impostazione e organizzazione anche di altre professioni: si dice, infatti - ed in parte è vero questo primo intervento del legislatore farà da battistrada anche per la disciplina e l'organizzazione di altre professioni. Sappiamo benissimo che esiste una concezione o una filosofia che è contraria, con argomentazioni rispettabilissime, all'organizzazione ordinistica della professione, in quanto vede in questo tipo di organizzazione l'espressione dello Stato autoritario che organizza anche il lavoro di professioni, ponendole sotto il controllo statuale. è però questa la sede, a mio parere, per affrontare tale tipo di discussione filosofica sul problema, avendo fatto ed operato un'opzione di fondo, ossia la scelta

su come, dopo oltre settant'anni, si intende organizzare, prevedere e disciplinare la professione di avvocato. Sono perfettamente convinto che,

Tutti noi siamo destinatari di quotidiani messaggi che criticano l'uno o l'altro aspetto del tipo di soluzione proposto.

tuttavia il legislatore ha l'onere di trovare una sintesi e una soluzione ai problemi sollevati.

nella sua espressione plenaria ma anche in sede di Comitato ristretto (presieduto e coordinato dal relatore, senatore Valentino), abbia evidentemente cercato l'interlocuzione con la categoria e le organizzazioni di categoria dell'avvocatura in plurime occasioni: il Consiglio nazionale forense, l'Associazione italiana dei giovani avvocati e l'Organismo unitario dell'avvocatura italiana sono stati all'evidenza interlocutori necessari in fase di consultazione e di audizioni. Non siamo stati insensibili ad alcuni suggerimenti,

Si è quasi rimproverata, invece, una posizione passiva della Commissione giustizia, che sarebbe stata quindi il «braccio armato» dell'avvocatura.

di superamento delle posizioni contrapposte, in una visione hegeliana della dialettica.

oggi la formazione dell'avvocato è modulata sulla patologia del sistema, in quanto la patologia si è così diffusa e sedimentata da diventare normalità. L'avvocato si forma sulla patologia; il sistema soffre l'avvocato si adegua al sistema, cercando di utilizzare tutti gli strumenti offerti per sfruttare la patologia. La visione che vorremmo avere è quella di pensare ad una avvocatura in un sistema normale,

Si pensi per un attimo come il fallimento del sistema processuale penale attuale sia

I riti alternativi gravano sull'avvocato, perché gli impongono una assunzione di responsabilità elevatissima. La responsabilità, però, presuppone preparazione, così come l'istituto della mediazione verso il quale andiamo nella riforma del processo civile significa preparazione, formazione. E allora, i punti che si è cercato di mettere a fuoco in questo disegno di legge sono: l'accesso, la formazione, il problema delle compatibilità, l'esercizio effettivo e il sistema tariffario. abbiamo inteso difendere il sistema tariffario minimo per tutelare la dignità di una professione e per evitare che le grandi *lobby* approfittassero della deregolamentazione per imporre prestazioni sottoremunerate.

attraverso la fase emendativa, possa migliorare la scelta e l'opzione proposta al Parlamento cui è approdata la Commissione giustizia. *(Applausi

fu soggetta ad alcune iniziative da parte di tutti gli schieramenti. Un *iter* lungo - ripeto - che ha visto una serie infinita di audizioni, incontri, verifiche

Certo, se abbandoniamo l'idea dei professionisti, del «serve ben altro», del «bisogna andare oltre», del «bisogna guardare gli scenari mondiali»,

dal 22 gennaio del 1934 al 2010, una parola, tenuto conto dei cambiamenti intercorsi, andava spesa. Se si ragiona su quello che oggi abbiamo davanti dobbiamo provare a individuare un punto di approdo e una possibile risposta agli apprezzamenti e alle critiche a questo testo.

gli Stati sono entrati nelle banche e hanno salvato le assicurazioni e che, di certo, in una crisi drammatica come questa ci sono state categorie, come gli artigiani e i liberi professionisti, che non hanno avuto

sono stati, cioè, i classici soggetti che interpretano l'autonomia, la libertà e l'esercizio di una professione o di una piccola impresa. Noi che siamo espressione

il senso di questa riforma? Ricordava prima benissimo il senatore Li Gotti alcuni punti qualificanti che sono stati oggetto di trattazione, sui quali si è intervenuto e su cui, rispetto ai testi originali, sono stati introdotti miglioramenti e modifiche. Mi riferisco

alla questione della specializzazione, invocata da tanti anni, all'inserimento dell'obbligatorietà dell'assicurazione del professionista

alla possibilità di iscriversi anche dopo i cinque anni dall'idoneità, così come sollecitato anche da alcune associazioni di giovani avvocati. Inoltre, rispetto

più volte evocato e sollecitato, ma io preferirei parlare di un'attenzione a chi si rivolge a un professionista,

e lasciata soltanto la possibilità di deroga ai massimi. Quindi, senza riprendere la discussione sul patto di quota-lite, che mi pare abbia trovato una soluzione definitiva nei lavori di Commissione, ritengo

di consulenza assai parziale possa scontrarsi con la possibilità di fare pratica; anzi, dovrebbe consentire a tutti quei giovani che non hanno le spalle coperte o studi professionali dietro

Signora Presidente, colleghi, non ho partecipato all'elaborazione del testo di questo disegno di legge, né al lavoro del Comitato ristretto; quindi, intervengo su questa

rispetto al ceto forense, cui appartengo ormai da oltre 30 anni.

Un prestigio che io vedo insidiato pesantemente, anzi - direi di più - compromesso ormai da molto tempo da alcune figure, se vogliamo stereotipi, stereotipi, che purtroppo corrispondono a molta parte della realtà di questa professione e che certamente non giovano, anzi pregiudicano gravemente la sua credibilità. innanzitutto lo stereotipo dell'azzeccagarbugli, dell'avvocato causidico

c'è la figura del professionista rapace, del rapporto professionale come trappola economica pericolosa per il cittadino e per l'utente. Questa è un'immagine dell'avvocato molto presente nella visione del cittadino comune, dell'uomo della strada; dobbiamo starci molto attenti e predisporre misure che tolgano spazio a questa figura. infine, l'immagine del ceto forense come casta, come gruppo chiuso, privilegiato, gerontocratico e impermeabile al nuovo,

Quale immagine dà in rapporto a quei tre stereotipi che nuocciono gravemente al al prestigio della professione? La mia impressione è che questo disegno di legge nuoccia gravemente sotto tutti e tre i profili, dal punto di vista di tutti e tre quegli stereotipi.

che dovrebbe caratterizzare il buon giurista, quel compito dal «Corpus iuris» di Giustiniano in poi dovrebbe essere quello di rendere il più possibile la formulazione della norma, di sfrondare la legge di tutto ciò che è superfluo e che, in quanto tale, genera incertezza ed è «sabbia negli ingranaggi». innanzitutto, che nella legge non si deve dare alcuno spazio a espressioni retoriche e prive di contenuto pratico. Questo ci insegnano i maestri del diritto.

«valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità delle persone»? Questa è una frase che, nel caso migliore, è priva di senso e, nel caso peggiore, dice invece qualcosa di profondamente sbagliato e cioè che l'ordinamento e il suo organo, che è l'Ordine degli avvocati, è lì per promuovere gli interessi economici della professione. Ma questo è compito di un sindacato o di un'associazione professionale; e da 60 anni a questa parte di sindacati unici imposti dalla legge in Italia non dovrebbero più essercene.

diffusione; la giusta causa di rivelazione, che è il cuore della norma, del contemperamento tra interesse alla conoscenza delle informazioni e interesse del singolo soggetto al segreto.

non rischiamo, sovrapponendovi una norma scritta oltretutto malissimo, che non fa onore alla competenza giuridica degli avvocati, di far sorgere gravi problemi di interpretazione? caso si sovrabbonda di espressioni vacue, retoriche e inutili, come quella che vincola l'avvocato alla «rigorosa» osservanza del segreto professionale. L'obbligo giuridico, o si adempie o non si adempie. È ovvio che l'adempimento debba sempre essere rigoroso. C'è un caso di verbosità inutile e retorica anche nell'articolo 7 dove,

Il giurista è chiaro, semplice. Il suo linguaggio è «sì, sì; no, no»; il «rigorosamente» e «solennemente» non sono termini che appartengono al suo linguaggio. Poi, Poi, sempre per rimanere su questo tema specifico, l'avvocato e i suoi collaboratori, dice il quarto comma dell'articolo 5 «non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie - questa idea della "specie" dei giudizi è nuova - su su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione». Ma nell'esercizio della professione si può anche venire a conoscenza del fatto che un gatto attraversa la strada o di altre notizie del tutto irrilevanti dal punto di vista dell'interesse al segreto. L'articolo 622 del codice penale definisce in modo molto preciso e rigoroso quali sono le notizie su cui l'avvocato può e deve rifiutare di deporre, ed è perciò esentato dall'obbligo di deporre in giudizio, dalle altre sulle quali questa esenzione non si come è formulata, autorizza l'avvocato a rifiutare di deporre su qualsiasi notizia, allargando a dismisura un'esenzione che non c'è alcun motivo di allargare, se non quello di allentare i doveri civili dell'avvocato, di creare un privilegio processuale al di là di ciò che è ragionevolmente proponibile. Veniamo al problema, forse il più rilevante dal punto di vista della tutela del prestigio della professione, di cancellare professione, di cancellare l'immagine del professionista rapace, del rapporto professionale come trappola economica pericolosa per il cittadino. cittadino. Oggi la situazione è questa. Il cittadino che si rivolge all'avvocato entra in un sistema di rapporti economico-professionali che per il cittadino stesso è pericoloso. Infatti, in caso di contrasto di interessi o di controversia su quanto sia dovuto all'avvocato come compenso per la sua opera, a giudicare di quel

questo è il dato da correggere, non da confermare o addirittura da consolidare, come viene confermato e consolidato nel disegno di legge un Ordine degli avvocati che sia posto prioritariamente non a tutela e promozione degli interessi economici della categoria - questa non può, non deve essere la funzione dell'ordine

tra l'avvocato e il suo cliente non può essere un organo composto soltanto da avvocati. È evidente che deve essere un organismo quantomeno composto pariteticamente da avvocati, magistrati e rappresentanti delle associazioni degli utenti, dei consumatori, dei cittadini. Questo è il minimo che come avvocati

che l'interesse economico del cliente. Se vogliamo liberarci di questa immagine ingiusta, che non corrisponde al modo di essere reale della stragrande maggioranza degli avvocati, dobbiamo dotarci di organismi preposti preposti a dirimere le controversie strutturati in modo da rispettare il principio di terzietà tra avvocato e cliente. cliente. La terza immagine negativa che grava sul nostro prestigio e della quale dobbiamo liberarci è quella del ceto forense come casta privilegiata, come categoria chiusa,

questa attività debba essere riservata soltanto a chi è iscritto all'albo degli avvocati? Mi dite un solo motivo per cui

assetto della disciplina va completamente riscritto, perché oggi noi abilitiamo a dare parere su dieci materie giuridiche diverse avvocati che sono competenti soltanto su una undicesima materia e sanno poco o niente di quelle altre dieci. a me per primo. Se mi chiedessero un parere in materia penalistica, tributaria o di diritto canonico, e se avessi l'ardire di accettare l'incarico e di fornire quel parere,

all'albo. Su questo terreno, quello dell'assistenza e consulenza stragiudiziale, lasciamo che siano i cittadini liberamente a scegliere di chi fidarsi; e anche chi vuole svolgere questa attività in modo professionale lasciamo che la possa svolgere: saranno i risultati di questa attività a dire se il suo consiglio è affidabile o non lo è. Questo è ciò che accade in tutti i campi del sapere umano; e deve poter avvenire

svolgere questa attività per il proprio datore di lavoro. Se questo è consentito nella forma del lavoro subordinato anche al non iscritto all'albo, perché mai non dovrebbe essere consentito di farlo in forma, che so, di consulenza coordinata e continuativa, piuttosto che libero-professionale? Abbiamo una grande ricchezza di dirigenti esperti in materia di diritto industriale, diritto dei brevetti,

di smettere di farlo in forma di dipendenti e cominciare a farlo aprendo uno studio di consulenza in materia di diritto internazionale, piuttosto che industriale o dei brevetti?

l'aggiunta di cavalli di Frisia contro l'accesso dei giovani. Addirittura è previsto l'esame di accesso al tirocinio. Vi è un incremento degli ostacoli che fa dell'accesso alla professione una gimcana difficile e sul piano burocratico; ostacoli formali prima ancora che sostanziali. Anche questo è profondamente sbagliato.

quel passaggio, evitando di porre un insieme di ostacoli intesi soltanto a rendere più difficile ai nostri figli di fare ciò che noi abbiamo potuto fare accedendo alla professione in modo molto più facile.

il metodo, caratterizzato da una scarsa volontà di ascolto su temi di rilevante importanza e soprattutto sul recepimento dell'ascolto. Oggi affrontiamo una discussione generale senza che sia ancora scaduto il termine di presentazione degli emendamenti che provvidenzialmente peraltro è stato prorogato fino alle ore 18 di venerdì prossimo, 16 aprile, dico provvidenzialmente perché la materia presenta particolari complessità e criticità. Inoltre, il ministro della giustizia Alfano ha convocato per oggi, 15 aprile, gli stati generali delle professioni. Malgrado non si conoscano ancora le intenzioni del Governo (il Ministro, a quello che capisco, verrà in Senato martedì prossimo), è prevedibile che la riforma della professione forense sottoposta già da ora all'Aula esemplifichi l'approccio del Governo alla questione delle professioni. In questo modo si vuole quindi estendere il metodo ad altre categorie professionali, così come riportano gli organi di stampa riferendo quanto annunziato dal Ministro della giustizia in vista degli stati generali convocati oggi, tesi, a quanto si capisce, a dare vita ad uno statuto generale delle professioni (cito al riguardo l'articolo del 13 aprile 2010 de oltre a notizie stampa, al momento non abbiamo ancora un intervento diretto del Ministro). Ebbene, comprendiamo benissimo che le liberalizzazioni non sono una priorità nell'agenda economica del Governo ma quello che non condividiamo è che si vogliano annullare i provvedimenti riformatori fatti in Italia negli ultimi quindici anni, che, devo dire, non sono stati nemmeno particolarmente stravolgenti della vita economica del Paese, ma che indubbiamente hanno portato degli effetti positivi. In sostanza, si va verso una controriforma dietro la quale la ragione politica è quella di accreditarsi come interlocutori di un'ampia categoria di professionisti che hanno problemi di agitazioni anche per motivi di sovraffollamento e che sono duramente colpiti dalla crisi. Quindi, con la riforma della professione forense si finirà con il dare un modello per le altre categorie con una giustificazione che è smentita dai contenuti della riforma stessa e dalle numerose critiche avanzate da più parti qualificate (non mi riferisco soltanto alle critiche dell'opposizione ma all'*Antitrust*, alle varie categorie di impresa, alle stesse categorie professionali degli avvocati, solo apparentemente riuniti in una volontà collettiva di approvazione di questo testo). La giustificazione sarebbe collegata alla difesa dei più deboli, soprattutto per quanto riguarda consumatori e giovani. Secondo gli economisti dell'*Antitrust*, le tariffe minime, punto focale di questa riforma, facilitano invece la collusione tra gli operatori e costituiscono una barriera all'entrata: due fattori che favoriscono chi è già nel mercato a scapito dei giovani

Il ministro Alfano, sempre secondo dichiarazioni di stampa, ha detto esplicitamente che l'abolizione delle tariffe minime ha danneggiato i professionisti italiani. Quindi, come giustamente rileva la stampa, per cementare il consenso si rilancia un modello corporativo basato basato su barriere all'entrata e vincoli di comportamenti. Domando e chiedo anche ai colleghi di maggioranza se proprio di questo il Paese ha bisogno. Fatta questa premessa, ritengo doveroso evidenziare, essendo stata una delle voci critiche contro questa riforma (che si è tradotta anche in emendamenti già presentati in Commissione e che intendo riproporre e approfondire per l'Aula con il contributo di altri colleghi del Gruppo del Partito Democratico, lo dico per chiarezza e coerenza), che il testo sottoposto alla Commissione giustizia nel suo complesso dopo la prima elaborazione del Comitato ristretto è stato poi fortemente rimaneggiato, anche in virtù di numerosi emendamenti che sono stati presentati dal Partito Democratico e dalle opposizioni. Il testo rispecchia in parte la proposta del Consiglio nazionale forense, ma, se possibile, per alcuni aspetti la peggiora. Tuttavia la filosofia di fondo che ispira la proposta di riforma della professione forense oggi alla nostra attenzione è sostanzialmente quella che molti anni fa ispirò la legge professionale, attualmente in vigore da oltre settant'anni. Quell'impianto è ancora ritenuto valido e la proposta di riforma rappresenta un blando tentativo di adeguarlo alle mutate condizioni sociali. Il risultato è una normativa che, se nel lessico può anche apparire moderna, come si è detto da parte di alcune associazioni di avvocati, con uno sforzo di fantasia, nella sostanza invece rimane permeata da una visione estremamente tradizionale e tradizionalista della professione di avvocato. Non so se sarà possibile con gli emendamenti ripercorrere la linea di un'intera riforma, ma certamente sarà possibile dare una linea chiara per il Partito Democratico. Democratico. Ciò che nell'immediato maggiormente richiamava l'attenzione dell'intera Commissione, quando è stato sottoposto il primo testo approvato, era prima di tutto la previsione e quindi l'accettazione di un potere regolamentare diffuso in capo al Consiglio nazionale forense, senza effettivi limiti, se non dal punto di vista formale e non sempre. La scelta di riservare questa potestà regolamentare al Consiglio nazionale forense era sostanzialmente motivata in un'ottica totalmente autoreferenziale.

quantomeno al Consiglio nazionale forense questo potere centrale e questa possibilità di emanare, con regolamento, una disciplina che finiva per integrare la legge e che non si capiva da quale fonte normativa potesse derivare. Tuttavia, se il potere regolamentare è stato in parte riportato, secondo il metro di norme e poteri, al Ministro della giustizia, il problema non è completamente risolto, anche dopo gli interventi modificativi. Un'altra norma che mi aveva profondamente colpito era quella che prevedeva che comunque il testo di questa riforma abolisse tutte le altre normative esistenti e avesse un carattere di specialità assoluta, che non avevo mai riscontrato in un atto normativo, anche perché le singole disposizioni che vengono abrogate devono essere coordinate. Sinceramente con questo sistema si poteva abrogare di tutto, perfino disposizioni importanti nell'ambito delle procedure penali, civili e amministrative, senza che si avesse la possibilità di intervenire. Dico questo per comprendere qual era addirittura il profilo iniziale rispetto al quale ci siamo confrontati.

anzi, di questa riforma credo non debbano essere contenti né i cittadini, né i giovani. Siccome noi dobbiamo stare con i giovani, come dice giustamente anche il presidente dell'*Antitrust*, perché sono anche il nostro futuro, su questo dobbiamo particolarmente investire. investire. Su questo primo punto credo dobbiamo essere fermissimi. È evidente che la giustizia richiede ammodernamenti e recupero di efficienza nell'interesse dei cittadini ed è quindi indispensabile che la riforma della professione forense sia parte della più complessiva riforma della giustizia. Con questo intendo dire che indubbiamente ci troviamo di fronte ad una riforma complessa, in cui le regole del mercato e della concorrenza, quindi le liberalizzazioni, devono essere comunque temperate anche in rapporto alla funzione che nel nostro ordinamento ha l'avvocatura, nel momento in cui viene chiamata a partecipare alla vita vita effettiva della giustizia. Vorrei ricordare che gli avvocati fanno parte dei Consigli giudiziari. Per chiarezza dirò che i Consigli giudiziari nelle sedi di corte d'appello, composti da

dunque parte del Consiglio generale della Corte di cassazione e soprattutto hanno una funzione pubblicistica che non può essere negata nel nostro sistema. L'attività difensiva, nell'ambito del processo penale, si svolge anche attraverso l'acquisizione di informazioni che gli avvocati possono ricavare dai testimoni

perché non possiamo prescindere da una valutazione congiunta dei due aspetti. Se non ricordo male, anche l'Unione delle camere penali, nel momento in cui ha svolto il suo congresso sulla riforma della giustizia penale, trattando il problema della riforma dell'avvocatura, ha

e consapevole del proprio ruolo, ciò non significa che non si debba investire sui giovani. In sostanza, l'avvocatura deve essere messa in grado di agire con elevata professionalità e competenza

garantendo il massimo di autonomia nell'esercizio del mandato, secondo gli indirizzi affermatisi nel diritto comunitario e nella giurisprudenza di Strasburgo e Lussemburgo che concepisce la professione forense quale servizio nell'interesse della collettività e dei singoli. Bisogna anche preparare questa libera professione così importante in maniera adeguata ad applicare le regole della concorrenza indicate dalle norme comunitarie, pur nel rispetto della deontologia e dell'offerta di un qualificato servizio per i cittadini. Questa riforma, dunque, deve contemperare molte esigenze, coordinare le nuove norme con la disciplina comunitaria, evitare che crescano i costi a carico dei cittadini nel ricorso alla giustizia, prevedere una disciplina innovativa nell'accesso alla professione che garantisca un'opportuna selezione dei molti aspiranti e un'adeguata formazione dei nuovi avvocati che consenta ai giovani di sviluppare le proprie capacità prevedendo la retribuzione dei praticanti durante il tirocinio e la partecipazione, possibilmente gratuita, ai corsi di preparazione, imporre poi un'elevata professionalità a tutti gli iscritti con un obbligo di costante aggiornamento attraverso strumenti, anche questa volta, possibilmente gratuiti. Credo che l'errore di fondo - mi sia consentito dirlo e l'ho detto più volte anche in Commissione ed il collega Valentino lo sa - sia stato quello di voler costruire ad un certo punto specularmente un Consiglio nazionale forense che fosse l'*alter ego* del Consiglio superiore della magistratura. Questa impostazione è assolutamente sbagliata perché il Consiglio superiore della magistratura è un organo di rilevanza costituzionale, ha delle altre funzioni, e perché il Consiglio nazionale forense, a differenza di quello che afferma, non è un organo di rilevanza costituzionale. Il Consiglio nazionale forense nasce con il regio decreto-legge n. 1578 del 1933 e sopravvive alla Costituzione perché la VI disposizione transitoria prevede che i giudici speciali possano sopravvivere alla Costituzione, peraltro, se vengono disciplinati con legge. Fino a questo momento non è stato fatto;

Tra l'altro, è veramente singolare che non soltanto si pensi di fare qualcosa di analogo al Consiglio superiore della magistratura, ma rispetto alla categoria della magistratura, che viene presa involontariamente come speculare, non si pensi di fare qualcosa di analogo. I corsi di formazione e la formazione dei magistrati sono gratuiti; esiste una scuola adesso presso il Consiglio superiore della magistratura che dovrà essere trasformata in scuola della magistratura. Tutto questo, invece, non viene calato nella realtà della riforma della professione forense, dove i corsi - mi dispiace dirlo dovranno diventare qualcosa che, non essendo purtroppo gratuiti e dovendo essere qualificati, darà anche adito ad un *business* economico su cui bisognerà stare molto attenti.

a questa asimmetria che si viene a determinare. Vogliamo dire che gli avvocati si devono qualificare come i magistrati? Tutti i magistrati, anche in Cassazione, anche il primo presidente della Cassazione, sono soggetti ad obbligo di formazione permanente; magari hanno una tale esperienza che ciò sembra quasi ridicolo, ma, in realtà, nessuno è escluso. Noi invece cosa prevediamo? L'accesso dei giovani ad una prova di preselezione per la pratica; l'impossibilità per i giovani di svolgere qualsiasi attività lavorativa mentre fanno pratica; l'impossibilità di essere pagati, quando questo era previsto perfino dal codice deontologico, per cui soltanto chi ha una certa consistenza economica ed anche familiare può

l'avvocato è titolare di diritti delegati dal proprio assistito e della sua difesa; la

di un'esigenza più generale di rivedere le normative sugli ordini professionali. Ho un approccio meno preoccupato, pur vivendo nella consapevolezza che

di opinione che speriamo possano essere ricondotte a sintesi quando tradurremo le nostre tesi in

tranquillo rispetto al dubbio e alla preoccupazione che sia un testo molto sbilanciato nel difendere le prerogative

questo di più credo non appartenga neppure alla consuetudine e alla generalità della produzione normativa di questo e dell'altro ramo del Parlamento. Si tratta

io l'ho immaginato così, e naturalmente ne chiedo conferma ai colleghi. Ho immaginato anche quel luogo come un ulteriore appello, come una prudenza, come un altro appuntamento, non inserito per appagare un bisogno e una preoccupazione, ma come un ulteriore effettivo esercizio che avverrà nella Commissione,

atteso che i regolamenti dovranno disciplinare buona parte delle materie, in quanto il testo è fatto di notevoli

assolutamente rivolta ad ampliare le prerogative corporative degli avvocati. Ci siamo messi al centro, come era giusto che fosse. E questo testo si pone proprio al centro nel tutelare gli interessi di una utenza - gli assistiti - che prima di ogni altra cosa debbono sapere di rivolgersi ad una categoria di professionisti che è in condizione di garantire qualità professionali e responsabilità nell'esercizio delle proprie funzioni.

funzione, la qualità del suo lavoro. È infatti dalla qualità del lavoro che discende un pezzo di buona giustizia anche nel nostro Paese. la formazione è centrale rispetto al testo, dove la troviamo come obbligo e non come

meritano e reclamano questo supplemento di impegno che per le altre categorie professionali non è stato messo in campo. Aspettiamo gli emendamenti;

anche il dibattito di ieri e di oggi ci servirà a tradurre in emendamenti più propri la nostre perplessità e le preoccupazioni che circondano il tema e il testo.

nei colleghi vi è l'auspicio che si possa giungere a un testo condiviso, perché sarebbe assai strano che su una materia come questa non si conseguisse l'obiettivo di una valutazione condivisa e di un testo comune, che naturalmente non vale soltanto per la categoria professionale degli avvocati: è infatti un tassello importante dell'intera riforma della giustizia e sarebbe quindi un bel preludio anche per il prosieguo di un dibattito che sulla giustizia appare complesso

e quindi l'approdo in Aula dello stesso, con una serie di contraddizioni che restano tali e sono difficili da affrontare

in considerazione della esigenza che il Governo e la maggioranza hanno avuto di dare qualche segnale in tema di riforma della giustizia. Ci si è detti che qualcosa bisognava fare:

e, quindi, all'arricchimento ed alle modifiche del testo che stiamo discutendo ed esaminando in quest'Aula. Rispetto a ciò, immaginare che il Parlamento e, segnatamente, la maggioranza

modo disorganizzato di procedere. Per questa ragione, noi abbiamo chiesto, non di rallentare l'esame del provvedimento, ma almeno di capire, una volta per tutte, quale sia l'opinione del Governo in materia. Questi sono alcuni limiti che ci portiamo dietro,

sia. L'avvocatura, infatti, svolge una funzione costituzionale: garantisce il diritto di difesa ed assolve, quindi, ad una funzione pubblica per la quale sono necessarie una qualificazione ed una specificità. Non partire da questo presupposto non significa mortificare le professioni, ma significa non dare attuazione piena ad un principio e ad un complesso di norme costituzionali che regolano il diritto di difesa e l'esercizio della giurisdizione, in quanto si sottrae alla garanzia dei diritti fondamentali e di libertà dei cittadini un pezzo importante dell'ordinamento. Quindi, l'idea che in questo settore la liberalizzazione debba travolgere tutto, anche la preparazione e la qualità del servizio e della prestazione professionale che si fornisce, è sbagliata ed è un'idea che non ci porta da nessuna parte. Certo, l'altro elemento che dobbiamo considerare, e che dal mio punto di vista sembra eccessivamente prevalente nel testo che stiamo esaminando, è quello della condizione economica del mercato dell'offerta forense. Sono

e non sempre - anzi quasi mai - ad una prestazione che viene remunerata in maniera eccessivamente bassa corrisponde una qualità costituzionalmente adeguata della prestazione forense. Queste sono le due questioni che devono essere affrontate. Dal nostro punto di vista, il testo che stiamo esaminando non fornisce una soluzione equilibrata rispetto a tali questioni. questioni. Credo che una prima considerazione vada fatta; l'hanno fatta la collega Della Monica ed altri colleghi, di maggioranza e opposizione, che sono intervenuti. Ci siamo sempre battuti per affermare il principio della centralità e dell'autonomia del Parlamento.

ma su richiesta, e non in via automatica o perché vi siano dei meccanismi legislativi che obblighino il Parlamento a scrivere le leggi sotto dettatura del CSM o delle associazioni di categoria dei magistrati. Se noi fino ad oggi - e lo dico ai colleghi di maggioranza - abbiamo abbiamo accettato e condiviso questo principio, esso deve valere per tutti, e anche per l'avvocatura. Non possiamo prevedere in questo testo che ogni atto di natura regolamentare...

del Consiglio nazionale forense. Questo organo deve essere sentito e deve essere l'interlocutore principale, insieme agli organismi rappresentativi dell'avvocatura, per il confronto a livello istituzionale nella produzione normativa dei regolamenti che sono funzionali ad una migliore organizzazione dell'attività dell'avvocatura; ma concedere o, anzi, ritenere che tutte le norme e tutte le regole debbano essere scritte al di fuori del Parlamento, riducendo l'organo legislativo a mera istanza di ratifica, mi sembra, proprio in ossequio a quel principio che invochiamo e applichiamo nel rapporto con la magistratura, magistratura, eccessivo e sbilanciato. Da questo punto di vista, è chiaro che il testo ci appare oltremodo squilibrato. Lo diceva anche il senatore Ichino prima: ci sono norme ridondanti che ripetono disposizioni che già esistono. È una sorta di testo unico ricognitivo, ma non credo che questo sposti molto sul piano della valutazione del testo. Mi preoccupa di più, ad esempio, la formulazione di alcune norme che, nel definire i principi cui devono ispirarsi alcuni regolamenti delegati (ad esempio, quelli che riguardano

con un intervento legislativo. Questa è materia che, al di là di principi generali, che bisogna fissare nella legge, deve essere affidata all'elasticità di un regolamento che possa anche tenere conto delle mutate condizioni condizioni economiche, culturali, istituzionali e sociali del tempo, che non determinano la necessità, sempre e comunque, di dover legiferare su questa materia. Credo che questo sia un aspetto, sia dal punto di vista metodologico sia dal punto di vista del merito delle questioni, che sarebbe opportuno apprezzare. Certo, c'è un problema che riguarda l'accesso alla professione. Capisco bene che, a fronte di 230.000 iscritti all'albo, quindi presunti avvocati, oggi gli organismi rappresentativi dell'avvocatura si trovino a dire che, poiché poiché la professione è diventata un ripiego per chi non trova collocazione nel mondo del lavoro con la laurea in giurisprudenza, un freno si deve porre. È un'osservazione giusta, dubito che il rimedio sia il migliore. L'idea di far pagare tutto questo ai giovani professionisti e ai giovani avvocati, senza che si faccia distinzione tra chi è meritevole e chi non lo è - perché il testo, da questo punto di vista, secondo me,

Né d'altro canto credo che stia in equilibrio il sistema relativo ai tirocinanti, nel momento in cui prevediamo un sistema di accesso e di selezione così rigido, così inutilmente rigido, a volte, da determinare poi il risultato che

anche questo potrebbe introdurre il tema del rapporto di lavoro subordinato, e quindi chissà che cosa, non possono svolgere alcun tipo di attività e debbono fare un minimo

non potendo lavorare né nel pubblico né nel privato, neanche *part-time*, per potersi mantenere alla formazione legale, dovendo fare la scuola di specializzazione forense, dovendo fare la formazione obbligatoria e così via, non so

un vantaggio, perché poi il rischio è che solo coloro i quali sono nelle condizioni economiche di poter fare questa scelta andranno avanti nell'attività professionale. Il giovane, quando esce dall'università, deve fare il *test* preselettivo anche se ha preso 110 e lode e quindi l'università l'ha già formato;

e di una selezione non sul merito ma sulle condizioni economiche, il che credo non consenta di valutare positivamente questo aspetto. Vorrei aggiungere poi, signora Presidente, che

se a questi praticanti non consentiamo di far parte dell'assemblea che elegge il Consiglio dell'Ordine o di far parte dei Consigli dell'Ordine, pur avendone ristretto il numero, e quindi non li coinvolgiamo nella conduzione dell'attività dell'avvocatura, ne facciamo una categoria a parte. Se questo è il senso, c'è un'incongruenza che va in qualche modo sanata.

per due ordini di ragioni. Innanzitutto perché, di fatto, i minimi tariffari sono stati sempre violati, nel senso che la prestazione è sempre stata oggetto di una pattuizione paralegale e paratariffaria, soprattutto per i giovani avvocati, e quindi alla fine non è cambiato molto. Questo vale anche al contrario, rispetto alla reintroduzione dei minimi tariffari. In secondo luogo, non credo che il tema della qualità della prestazione, della minore onerosità della prestazione e del favore nei confronti del cliente

cosa che non viene mai fatta. Non ho mai trovato nella mia attività professionale una sentenza che nel liquidare le spese giudiziali abbia mai rispettato il tariffario. Certamente

sono stati eliminati. Un'ultima considerazione e concludo.

fatto che nel provvedimento sia contenuto un complesso di disposizioni normative che disciplinano l'ordinamento forense che risale a poco dopo il primo dopoguerra.

Pertanto, il ruolo sociale che riveste non può essere lasciato alla mercé del mercato. Mi sfugge chi dei colleghi, per esempio, ha detto che nelle audizioni

la funzione istituzionale dell'*Antitrust*, del garante del mercato, è quella di basare tutto sulla massima concorrenza, pertanto sui prezzi più bassi che la concorrenza spietata o più larga possibile consente: ma noi vogliamo fare della giustizia un mercato libero? Mi Mi sembra che dagli interventi anche dei critici sia emersa la necessità di una grossa professionalizzazione, di una grossa formazione, cioè di una garanzia per il cittadino di mettere in mano (perché di questo si tratta) la propria vita a persone che la sappiano gestire al meglio.

una visione rispettabile, ma vorrei giocare su questo aspetto: chi dei radicali, dovendosi costruire una casa, penserebbe di mettersi in mano al primo che afferma di essere in grado di costruirla

sistema costituito, normato e regolamentato, otteniamo anche la massima garanzia da parte di chi, incapace in qualsiasi settore di provvedere in modo autonomo, si deve chiaramente mettere in buone mani.

gli esami di Stato; possiamo pensare che l'esame di Stato potrebbe anche non servire. A questo punto, immediatamente, ci sarebbero circa 100.000 avvocati all'anno in più; cancelliamo anche i limiti tariffari e lasciamo che tutto venga regolato dal mercato; cancelliamo anche l'Ordine, perché non avrebbe più senso. Chiunque, dotato di media ponderazione, direbbe che qui si rischia di cadere in una giungla, e mi sembra che nessuno lo voglia.

Se vogliamo, critichiamo come il tirocinio viene gestito e normato ancora oggi, lasciato alla libera interpretazione di tanti professionisti,

Ho letto, invece, alcune interessanti innovazioni nel nuovo testo che si propone all'Assemblea;

di attività. Tra l'altro, la specialità non diventerà una riserva di attività, altrimenti questa sarebbe un'altra limitazione

la difesa d'ufficio bisognerà avere la specialistica in diritto penale. La seconda innovazione importante riguarda la sicurezza che si dà all'esterno, con l'obbligo per il professionista di assicurare, come fanno tanti altri professionisti, la propria attività.

Sembrava che le problematiche della disoccupazione giovanile dovessero crollare in un unico momento, in un sol frangente, eliminando tutte le croste, i limiti e i vincoli.

le buste chiuse con i limiti minimi, in cui è la stessa amministrazione che dice: «Tu non puoi darmi quello che ti chiedo sotto una certa soglia, perché altrimenti so già che mi darai qualcosa che non è quello che ti sto chiedendo e che ci sarà qualcosa che

Il professionista può anche decidere di erogare la prestazione, in termini volontari, per giustificati motivi, non solo sotto il minimo, ma addirittura a titolo gratuito. Questo non lo si vieta e non lo si limita, anzi lo si prevede addirittura per legge.

proficuo impegno. Ci sembra che ciò vada sempre nella direzione di pretendere maggior serietà e professionalità da parte del professionista. Vado a chiudere. Se i fini di questa la qualità della prestazione, la responsabilità e la formazione degli operatori in quanto garanzia della difesa, garanzia di un bene di un bene alieno all'ordinamento forense, ma proprio di chi a questo si rivolge, io dico che questa norma è una buona norma, raggiunge fini e obiettivi lodevoli. Sarà un documento perfettibile (vedremo gli emendamenti in che direzione andranno), ma

anche perché chi di noi è abituato a «dirla direttamente» in questo caso la manderebbe a dire. Di solito si dice «io non la mando a dire», mentre qui dovrei farlo perché perché anche coloro che sono intervenuti hanno preso i loro bagagli e se ne sono andati. Io invece ho ascoltato tutti, anche ieri sera benché non dovessi intervenire. Ora però, proprio per la natura, diciamo, estemporanea e anche perché io sarei chiamato a parlare per il Gruppo di maggioranza relativa su questo argomento, dato che abbiamo ascoltato molti discorsi sostanziosi e coloriti, io ho il dovere, più che il diritto,